2007 Presidente del Consiglio dei ministri Ministro trasporti (Governo Prodi-II) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2007, n.117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione